Il senso di questa discussione si riassume in tre punti molto precisi: il nostro Paese spende troppo, siamo indebitati oltremisura e non cresciamo. Questi sono i tre assunti che si ricavano dalla Decisione di finanza pubblica presentata che con questo documento certifica in qualche modo il fallimento di una politica: un fallimento ormai sotto gli occhi di tutti.

il Governo non predispone nessuna terapia di intervento, nessuna terapia d'urto. È davvero impressionante come di fronte ad alcuni dati, come ad esempio quelli del debito,

ieri è stato certificato dalla Banca d'Italia che il nostro debito ammonta a 1.843 miliardi

non si preannuncia una strategia di intervento;

Ricordo che sono 100 i miliardi di evasione all'anno. Francia e Germania stanno mettendo a punto una loro strategia comune per una riforma fiscale nei loro Paesi che sia uniforme

La prima cosa da fare, se vogliamo anche incentivare i nostri ragazzi a studiare per davvero e a premiare il merito - come voi dite sempre e non fate

i nostri cittadini cominceranno guardarci in faccia.

Ciò mi preoccupa anche in relazione a quanto avvenuto ieri alla Camera dove, di fatto, è stata bloccata la riforma dell'università

però ben quattro condizioni che mi preme ricordare: integrare il fondo per l'offerta formativa delle scuole; ripristinare le dotazioni del fondo di finanziamento ordinario dell'università; coprire l'eliminazione del blocco degli scatti di anzianità per il personale della scuola; estendere l'eliminazione del blocco degli scatti di anzianità per i professori ricercatori universitari. riguardo fornire qualche dato perché ci si renda conto di quale sia la situazione in particolare dell'università italiana, ma anche della scuola italiana.

Per quanto riguarda l'anno accademico 2010-2011, vi è un taglio complessivo del 20 per cento dei corsi di laurea. Queste due

numero di studenti è inferiore alla media OCSE. È arrivato il momento di tornare ad investire risorse nel settore dell'istruzione e della ricerca, perché altrimenti il nostro Paese non sarà competitivo. Se la Germania cresce più di tre volte rispetto all'Italia

per uscire da questa situazione di crisi. Tale mancanza di strategie e di linee programmatiche e di sviluppo è riscontrabile anche per quanto riguarda il sistema salute del nostro Paese. Non se ne parla nello schema di Decisione di finanza pubblica, se non per alcuni cenni in pochissime righe. Eppure, il sistema salute è una voce importante della spesa pubblica. inoltre sottolineare, signora Presidente, perché si tratta di un dato molto trascurato, che esso ha come indotto un sistema produttivo di ricerca e di innovazione nel campo dei farmaci, dei dispositivi medici e della strumentazione diagnostica

Questo sistema è oggi messo a dura prova da cambiamenti profondi, che si definiscono su alcuni fattori. Vorrei citarne alcuni: quello epidemiologico, l'aumento delle aspettative di vita, il conseguente aumento esponenziale delle malattie croniche, cronico-degenerative ed oncologiche. Questi mutamenti richiedono un sistema di cure sempre più raffinato ed innovativo: pensiamo solo all'uso delle particelle dell'atomo nella cura delle malattie oncologiche. Si tratta di cure che si devono sviluppare in un tempo di vita lungo, quale è stato conquistato proprio grazie alle innovazioni in campo scientifico. altro settore di cambiamento che ha interessato la sanità è rappresentato dalla modifica del Titolo V della Costituzione, che ha fatto sì che le prove di federalismo di cui ci si riempie continuamente la bocca nel nostro Paese siano proprio state fatte sul sistema sanitario. In questi anni è stato tra l'altro inaugurato un sistema pattizio tra Stato e Regioni, che ha significato cambiare profondamente un modello che si basava sui ripiani a piè di lista, per approdare ad un sistema di risorse programmate e ad una forte responsabilizzazione delle Regioni nella spesa. Questo cambiamento epocale ha dato dei frutti: vi sono esempio Regioni virtuose, ma vi sono anche Regioni che sono state in qualche modo obbligate, perché avevano accumulato un forte debito, a predisporre dei piani di rientro e a rientrare rispetto al debito accumulato. Per questo abbiamo ritenuto grave lo strappo istituzionale fatto con il taglio unilaterale che si è consumato con la manovra di giugno e che viene ribadito nel documento oggi in discussione. A fronte A fronte di tutti questi cambiamenti, abbiamo sperato che nel documento ci fosse una valutazione del Governo e del Ministro competente, anche per comprendere dove si vuole andare con il sistema salute. Va considerato che ormai entriamo in Europa in modo sostanziale, e nella prossima sessione di bilancio europea ciò sarà ancora più evidente. Il documento al nostro esame poteva essere l'occasione per misurarsi sulle prospettive della sanità italiana, che oltre tutto deve commisurarsi sempre più con un sistema salute europeo competitivo, perché altri Paesi, ad esempio la Francia, investono più di noi nella ricerca e nell'innovazione. Probabilmente non se ne sono ancora accorti tutti a sufficienza, ma c'è molta gente che va a curarsi in altri Paesi europei, come la Spagna o la Francia; questo succederà sempre più spesso, se anche noi non investiremo con più forza nel sistema della ricerca e dell'innovazione in campo sanitario. Noi però sappiamo che tutto ciò che stiamo dicendo non è trattato nei documenti ufficiali. Il ministro Sacconi, ad esempio, a proposito del federalismo, in un'importante rivista politica ha detto che federalismo significa sapere far di conto (*ergo*, occorre tagliare la spesa) e che lo Stato deve essere un agente terzo ed imparziale rispetto al cittadino e ai produttori di servizi, che il Ministro tra l'altro mette sullo stesso piano, siano essi pubblici, privati, *profit*, *no profit*. Questo modo di intendere il federalismo è inaccettabile, come è inaccettabile tagliare le risorse senza tenere conto dei LEA, come ci hanno ricordato tutti i presidenti delle Regioni, indipendentemente dalla loro collocazione politica. È ugualmente inaccettabile l'idea che il principio di sussidiarietà venga applicato unicamente non solo per ridurre la presenza del pubblico nella produzione dei servizi, ma anche per deresponsabilizzare le istituzioni rispetto a una garanzia che deve essere data

ha investito 940 miliardi di euro in dieci anni, in un Paese in cui tra l'altro si è sempre puntato sulla sanità privata e che ha un sistema che incide il doppio del nostro sul prodotto interno lordo. documento in discussione nulla si dice dei costi standard, che possono essere applicati cambiando radicalmente in un modo o nell'altro, positivo o negativo, il sistema della sanità e i rapporti tra le Regioni che stanno al Nord e al Sud. Si tratta di una questione particolarmente complessa, perché è difficile conciliare conciliare l'efficienza della spesa con la sua efficacia, con i LEA ed anche con degli obiettivi-salute. Vogliamo dunque chiederci quali sono gli obiettivi-salute che questo Governo ha per il nostro Paese? I tagli lineari apportati a giugno sulla sanità

verranno affrontati la riduzione di risorse nella formazione del personale, l'aumento del precariato, l'invecchiamento del personale medico (presto si ridurrà notevolmente il numero dei medici), la mancanza di alcune figure specializzate

e privo di contenuti significativi ed in qualche modo disattende lo spirito della legge 31 dicembre 2009, n. 196, visto che si limita a registrare la situazione attuale e gli andamenti previsti per il triennio,

abbiamo davanti, confrontandoli con gli utili contributi pervenuti dalle audizioni. Ma ciò che dimostra tutta la debolezza dell'azione di Governo è l'assenza delle informazioni previste dall'articolo 7 della legge sulla contabilità che riguardano gli obiettivi sul terreno della crescita economica. Non si intravede alcun cenno sulle strategie per uscire dalla grave crisi e per recuperare la capacità competitiva del Paese. Si potrebbe dire lo stesso per la mancata presentazione delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica, come detta l'articolo 10 della stessa legge, al fine di coinvolgere in questo processo non solo il Parlamento, ma anche le autonomie locali. Ci preoccupa inoltre il comportamento del Governo anche rispetto ai nuovi passaggi che dovrà affrontare per adempiere alla prossima riforma della politica economica europea, in particolare per adeguarsi alla nuova sessione di bilancio europeo. Ma non è parlando di questioni di forma e di metodo che intendo continuare questo intervento; esse non interessano nessuno e nemmeno sono di qualche utilità per tutti quei cittadini che continuano a pagare in prima persona gli effetti negativi della grave Per essi non si intravede uno spiraglio, un filo di speranza per il futuro. Nonostante le tante promesse e i toni rassicuranti dei vari ministri, i dati reali ci mostrano un Paese che arranca, molto più degli altri paesi europei. Basti leggere il decimo rapporto Caritas - Fondazione Zancan, dal quale emerge che i poveri in Italia sono 8.370.000. Contrariamente agli altri Paesi europei, da noi più alto è il numero dei figli, maggiore è il rischio povertà. I dati riportati ci dicono ancora che la povertà si conferma un fenomeno del Sud, delle famiglie numerose o monogenitoriali e di chi ha bassi livelli di istruzione. Mi soffermo su altri due aspetti, che in qualche misura denotano tali difficoltà: il mercato del lavoro ed i consumi. È da qui che è necessario partire. Non è un caso che il Partito Democratico abbia posto con forza in questi due anni due richieste semplici, ma fondamentali: la riduzione della pressione fiscale per i redditi medio-bassi, cioè i redditi da lavoro dipendente e da pensioni, attraverso l'innalzamento delle detrazioni d'imposta, ed interventi per la ripresa dell'occupazione, attraverso misure di tipo fiscale e infrastrutturale. Il Governo si è sempre trincerato dietro il convincimento che nei momenti di crisi non si può mettere mano alle riforme. Adesso, però, non è la maggiore forza di opposizione a chiederlo; è l'Unione europea a prevedere il Piano nazionale di riforma. Con quali proposte si presenterà a questo appuntamento di novembre il Governo italiano? Noi vorremmo perlomeno discuterne. Tornando ai problemi sopraesposti, ripropongo alcuni dati che emergono dal documento: il tasso di disoccupazione si attesta all'8,2 per cento, livello che rimane tale fino al 2011; solo con il 2012 si intravede un lieve miglioramento. Tralascio i dati relativi alla cassa integrazione guadagni, che però ci devono fare riflettere soprattutto per quanto riguarda i 225 milioni di ore di cassa integrazione in deroga. Ma c'è un dato sul quale non si può soprassedere, cioè la disoccupazione giovanile, che è secondo l'ISTAT al 25,9 per cento. Si tratta di un vero dramma nazionale, che mette a repentaglio il futuro dell'Italia, perché si sta bruciando un'intera generazione, si stanno sprecando tante risorse umane e tante competenze, si sta minando la futura classe dirigente del Paese. Questa è la vera emergenza, ma la DFP non prevede alcuna misura per invertire tale tendenza. C'è poi il tema della partecipazione delle donne alla vita produttiva. L'ultimo «*Global gender gap report*» stilato dal *World Economic Forum* classifica il nostro Paese al 74o posto tra 134 Paesi presi in considerazione, scavalcato quest'anno da Ghana e Malawi. Questa pessima *performance* è dovuta soprattutto alle difficoltà per le donne nell'accesso al mondo del lavoro e alle minori opportunità. Parlando di sviluppo economico, va ricordato che il recente studio della Goldman Sachs ha calcolato che, se in Italia le donne partecipassero al mercato del lavoro nella stessa misura degli uomini, il nostro prodotto interno lordo crescerebbe del 13 per cento. Non elencherò le nostre proposte; esse sono contenute nella proposta di risoluzione alternativa del PD e riguardano misure concrete e cantierabili, che spesso in quest'Aula abbiamo illustrato. In conclusione, questo Governo continua ad andare avanti senza ascoltare né l'opposizione né i vari attori sociali né il disagio sempre crescente dei cittadini. «*The* *show must go on*», si dice, a prescindere. Onorevoli colleghi, noi del Partito Democratico, e con noi tanti italiani, auspichiamo che questo spettacolo finisca quanto prima, a beneficio dell'intero Paese.

Il Governo ha fatto conoscere la propria intenzione di accettare la proposta di risoluzione n. 5, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125-*bis*, comma 4, ultimo periodo, del Regolamento. questo momento decorre pertanto il termine di un'ora a disposizione dei Gruppi per avanzare proposte emendative sul testo della proposta di risoluzione n. 5.

Signora Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, nello svolgere una riflessione ragionata sullo schema di Decisione di finanza pubblica presentato dal Governo per gli anni 2011-2013, vorrei sottolineare soprattutto i dati positivi riscontrati che, seppur in misura contenuta, costituiscono segnali significativi di una prospettiva di ripresa dell'economia mondiale, di quella europea e, in particolare, di quella del nostro Paese.

e, dunque, dei diversi momenti di definizione programmatica dei Paesi membri dell'Unione. È una riforma molto attesa che costituisce un progresso significativo nella costruzione di una *governance* europea e nel rilancio del ruolo dell'Unione nel panorama economico mondiale. Già nel prossimo novembre saremo, quindi, chiamati a presentare la bozza del piano nazionale di riforma, in coerenza con il nuovo schema europeo, sul quale si concentrerà la discussione politica economica a livello comunitario. I dati che emergono dal documento in esame mettono in luce che il miglioramento delle condizioni economiche mondiali si sta consolidando, grazie soprattutto alle eccezionali misure di stimolo monetario e fiscale adottate dai Governi in ambito internazionale; misure ingenti che, sebbene abbiano comportato riflessi di sacrificio e di rigore nella comunità civile, sono risultate decisive per un'evoluzione positiva della crisi globale. Nei primi due trimestri del 2010 l'economia mondiale è cresciuta - in linea con essa, anche la *performance* dell'area euro, trainata dagli apprezzabili risultati dell'economia tedesca - e ha registrato un miglioramento in termini di crescita del PIL dell'uno Molti Paesi europei, in questi mesi, hanno adottato e continuano ad annunciare politiche di consolidamento fiscale per assicurare la sostenibilità del debito pubblico e, sebbene in misura differenziata e con prospettive non esaltanti, gli attuali piani di risanamento dei conti pubblici sembrano andare nella giusta direzione. Non si può, quindi, non prendere atto che le misure di riduzione del deficit adottate da questo Governo - che hanno imposto rigore e austerità - hanno, in pari tempo, condotto a risultati che progressivamente ripagheranno i sacrifici richiesti al nostro Paese. Nel secondo trimestre la ripresa in Italia si è rafforzata e, come affermato anche dal ministro Tremonti, la crescita proseguirà, seppure a velocità ridotta, anche nella seconda parte dell'anno. Persiste, senza dubbio, un problema di competitività che ha limitato la crescita delle esportazioni, ma la rinnovata espansione del commercio mondiale ed il deprezzamento dell'euro consentono di formulare una previsione positiva per l'Italia, protesa verso un recupero ed un miglioramento dell'*export*, a sostegno della futura crescita. vorrei ricordare l'impegno che il nostro Governo ha profuso a favore del *made in Italy* e gli interventi normativi a tutela del marchio italiano, per garantirne una maggiore trasparenza e tracciabilità a favore di una maggiore competitività industriale e produttiva. Nonostante la violenza della crisi, quindi, i risultati che emergono evidenziano la tenuta complessiva del sistema Paese, che consente di esprimere un giudizio di adeguatezza sulle misure messe in campo dal Governo per fronteggiare il difficile momento di congiuntura economica. Anche le condizioni delle imprese sono migliorate, sostenute dal recupero della produzione industriale, degli ordinativi, dei fatturati e della fiducia. Si tratta di un giudizio positivo che fornisce indicatori in favore di un buon andamento della produttività anche nei prossimi mesi. Rispetto alle stime contenute nella dello scorso maggio, lo scenario appare più favorevole. Si è registrata infatti una revisione al rialzo della crescita attesa per il 2010, nella misura dello 0,2 per cento, ed una revisione al ribasso di pari entità per il 2011. Bisogna anche dire che sulla dinamica dei tassi, molto importante per il nostro Paese, ci sono condizioni migliorative rispetto alla RUEF. Coniugare la stabilità delle finanze pubbliche con la necessità di non deprimere la ripresa economica resta, dunque, la sfida maggiore sullo scenario mondiale e l'obiettivo primario per la nostra economia nazionale nei prossimi due-tre anni. Ma, seppur nella consapevolezza di dover proseguire ancora verso una politica di responsabilità, è necessario scorgere nell'azione di Governo quei segnali positivi che costituiscono un incoraggiamento ai mercati e alla fiducia degli attori che in esso operano. Non si può non considerare che la *performance* dell'Italia durante la crisi abbia dimostrato, per le sue caratteristiche strutturali, più solidità e meno vulnerabilità rispetto ad altre economie avanzate; il nostro sistema bancario è rimasto in gran parte immune dalle turbolenze internazionali ed anche il settore immobiliare è stato colpito solo marginalmente dagli squilibri mondiali. Occorre rilevare che, come è auspicabile, se venisse accolto dall'Unione europea quel criterio di valutazione del debito che apprezza il dato aggregato, il valore del debito pubblico sommato a quello privato, collocherebbe l'Italia tra i Paesi "in sicurezza", consentendo anche politiche più espansive di sostegno alle famiglie ed alle imprese. D'altro canto, l'Italia sconta oggi la debolezza strutturale e l'ingente debito pubblico risalenti ad un periodo antecedente al dispiegarsi degli effetti della crisi globale. Sebbene il *trend* per l'economia italiana si ponga in linea con quanto atteso per gli altri Paesi europei, le cause dei suoi minori margini di crescita e di una velocità di recupero più lenta, rispetto alla media europea ed alla Germania in particolare, non possono ricercarsi in fattori o mancanze imputabili a questa compagine istituzionale, ma devono necessariamente collegarsi alle diverse peculiarità strutturali italiane, alle condizioni pre-crisi, che scontano un divario nella produttività, nelle infrastrutture, nei servizi accumulato, storicamente, in decenni. Fatalmente ed inevitabilmente, quindi, le criticità strutturali di crescita dell'economia italiana hanno trovato il loro riflesso nell'attuale fase congiunturale e, conseguentemente, nelle prospettive di ripresa e di uscita dalla crisi. Vorrei sottolineare quanto sensibilmente, in Italia, incidono sull'economia la carenza di fonti primarie di energia e la riduzione della disponibilità energetica negli ultimi anni. La diminuzione delle importazioni di petrolio e di gas naturale è quindi un obiettivo primario che questo Governo si prefigge di realizzare, proseguendo sulla strada della riforma del settore, in una prospettiva di sostenibilità, che sappia, sì, favorire la concorrenza e l'apertura dei mercati, ma che riduca i costi a carico dei consumatori e limiti l'impatto sull'ambiente. In quest'ottica deve inquadrarsi la scelta del Governo di riavviare parte della produzione di energia elettrica da fonte nucleare; una scelta che, peraltro, potrà sviluppare i suoi effetti positivi e soddisfare parte del fabbisogno energetico solo nel medio-lungo periodo. Appare allora quanto mai necessario puntare sul rilancio degli investimenti, incentivando il sostegno alle imprese, riducendo le rigide maglie della burocrazia e proseguendo sulla strada del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione. Una sfida, in sintesi, all'Italia di rafforzare l'azione di risanamento del bilancio e di concorrere, dinamicamente, al consolidamento di quella strategia di sviluppo europeo che, sola, consentirà all'Unione di partecipare ai processi decisionali globali.

mi chiedo quale utilità reale possa avere lo schema di Decisione di finanza pubblica se non riempie di contenuti, come diceva il relatore di minoranza, senatore Morando, le proprie previsioni; se addirittura ne autoriduce la portata, dichiarandolo superato dalla manovra di luglio; se ne dichiara l'inutilità vista la sessione di bilancio europeo, in un incredibile atteggiamento di attesa, anziché di partecipazione, di protagonismo, di occasione di confronto in se non dice, per esempio, su quali settori, con quali strategie, si pensa di rimuovere gli ostacoli che impediscono un'adeguata crescita. Il grande problema di questo Paese è che da troppo tempo è in affanno. Una previsione del tutto virtuale, con numeri sospesi nel vuoto, rende tutto il non senso di questa discussione. Credo che questo Paese, sfiduciato e disilluso, possa riprendere speranza solo se avverte in chi lo guida un approccio onesto, trasparente e molto concreto.

(una volontà soprattutto di progettazione del cambiamento, e non di improvvisazione, di *spot*, come usa fare questo Governo); in secondo luogo, quali sono le sue potenzialità, i suoi punti di forza, quali sono le vocazioni su cui investire e gli spazi per competere nel mondo. Noi, signora Presidente, abbiamo un settore, l'agroalimentare, che rappresenta entrambe queste condizioni, fino ad assumere livelli di paradosso. È un settore che contiene tutte le criticità, che una crisi senza precedenti ha messo a nudo ulteriormente; una crisi che ha colpito il Sud come il Nord e che ha evidenziato quanto sia urgente ed indispensabile una riconversione profonda di carattere strutturale, e non altro. Per contro, è uno dei settori con maggiori prospettive, che presenta spazi e opportunità già oggi, che bisogna però conquistarsi e cercare. Le criticità sono sintetizzate nei numeri. Il numero uno dei problemi è l'emergenza ricambio generazionale: solo il 7 per cento delle imprese agricole è nelle mani di un quarantenne o con qualche anno di meno; ben il 44 per cento, cioè quasi la metà delle imprese, è in mano ad

degli imprenditori che stanno cedendo la proprietà a forti soggetti commerciali, molte volte stranieri, per diventarne dipendenti o contoterzisti. In altre parole, un fenomeno in cui si cede direzione d'impresa, saperi, *know-how* in mano ad altri. È la resa dei produttori; è l'Italia agricola che si assesta ad un livello più basso e che rinuncia alla sfida e al rilancio. Soprattutto è alto il rischio di un *made in Italy* agroalimentare che, diminuendo la produzione in Italia, si trasforma in piattaforma di stoccaggio, di sola trasformazione, di passaggio, svendendo l'unico patrimonio non replicabile e non localizzabile. Il paradosso è proprio questo: una grandissima difficoltà a competere, fuori e dentro i confini nazionali, con un prodotto che è riconosciuto nel mondo: una difficoltà che si registra mentre cresce la domanda di alimenti, semplicemente per la rapida crescita demografica, che induce più domanda di cibo (dovrà crescere la possibilità di accesso al cibo da parte di chi oggi ne è scandalosamente escluso) cresce la domanda di prodotti di qualità alta; crescono nel mondo coloro che possono accedere al prodotto di qualità alta. In un mondo globale che tutto omologa, cresce poi la domanda di autenticità; cosa esiste di più autentico di un prodotto e del suo territorio insieme? Un prodotto integrato, tutto ancora da scoprire e da proiettare sui nuovi mercati. L'agroalimentare dunque è un settore destinato all'espansione sia quantitativa, che qualitativa. Perché allora non riusciamo a cogliere questa opportunità? In primo luogo perché il nostro settore è troppo frammentato, non ha sufficiente organizzazione per andare a proporsi sui nuovi mercati, perché è appesantito da inutili burocrazie, che spesso supercontrollano le questioni formali e non vedono la sostanza. Non si affronta con coraggio quell'inefficienza dentro la catena alimentare che moltiplica i costi dei prodotti senza aumentare il loro valore reale, indebolendo reddito e autonomia dei produttori, penalizzando i consumatori, spinti alla ricerca del minore costo senza garanzie, qualità e trasparenza. In secondo un Governo che, anziché fare dichiarazioni, credesse davvero nella vocazione agricola di questo Paese come uno dei settori strategici in cui si può giocare la modernizzazione e il futuro. Servirebbe un Governo determinato ad andare in Europa a sostenere una riforma della PAC rivolta al futuro; che governi e non subisca le evoluzioni; che premi i comportamenti virtuosi e non lo *status*, le inerzie legate alla proprietà e alle rendite;

e orienti in questa visione l'Europa; che contempli nuovi indicatori assieme alle efficienze aziendali, alle efficienze dei sistemi, alle razionalità logistiche; che contempli il valore del cibo come valore primario e l'ecosostenibilità come nuova frontiera della competizione, il valore del consumatore e la sua salute al centro, l'agricoltura come valore pubblico di un territorio, di una comunità, ma non nel senso di assistenza passiva ma come nuova visione di competitività. Questo è il Questo è il futuro che dovremmo essere capaci a mio avviso di disegnare oggi, per attrarre giovani e nuove professioni, per individuare nuovi percorsi formativi per un settore che, dentro una parola arcaica, contiene il più alto tasso di potenziale di modernità. Siamo lontani anni luce da tutto a questo.

- come diceva bene il collega Andria - il minimo per affrontare l'emergenza. Nulla sulle emergenze climatiche, sul costo del lavoro e su sostegno e costi di produzione. Neppure una parola sulla PAC. In questi In questi mesi un dibattito ha coinvolto l'Europa: non si è dedicata una sola ora alla revisione del bilancio europeo della PAC. In compenso, rimarrà alla storia, in capo a questo Governo, l'indimenticabile questione delle quote-latte. Questo Paese, l'Italia del*made in Italy,* merita veramente qualcosa di diverso: di veramente molto diverso.

con documenti alla mano - di interpretare il pensiero dell'intera Commissione, indipendentemente dal coraggio di ammettere alcune realtà. L'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 prevede che la Decisione di finanza pubblica debba, tra l'altro, individuare, oltre agli obiettivi di natura economica, anche quelli programmatici dei saldi e del debito. sul settore scuola, università e formazione, caro Vice Ministro, cara relatrice, non c'è nulla. Lo dice lo stesso presidente della 7a Commissione, senatore Possa, quando testualmente afferma che nello schema «non ci sono elementi di diretto interesse della Commissione, a parte i dati contenuti nella tavola 2.10». In quella tavola, al sesto rigo del Capo III, è scritto «Blocco automatismi stipendiali 2010-2011-2012-Comparto scuola», con economie rispettivamente di 320, 640 e 960 milioni di euro. Questo è l'unico riferimento alla scuola che un grande Paese europeo come l'Italia fa nella sua programmazione finanziaria. Se pensiamo ai traguardi e alle idee condivise che i Paesi europei hanno fatto propri a Lisbona ci rendiamo conto di essere fuori da quell'alveo e assai lontani dalla convinzione che puntare sulla formazione e sulla ricerca significhi alimentare la crescita complessiva anche economica di un Paese, soprattutto di un Paese come l'Italia che, come spesso ripete il Ministro plenipotenziario dell'economia - ma non è solo dell'economia, ormai è di tutti i Dicasteri - ha essenzialmente problemi di crescita. Non è un caso se la Francia, nonostante la crisi economica, non tocchi i fondi destinati a scuola e università e se la più lungimirante Germania, nonostante una durissima manovra finanziaria che taglia 100 miliardi di euro in quattro anni, stanzi circa 11 miliardi in più per formazione e ricerca. Ma quello che più sconcerta è che il contenuto del documento in esame contraddice palesemente quanto affermato in quest'Aula - e non solo - dal Governo. Il 29 luglio 2010 il ministro Gelmini affermava

mai di ciò non vi è traccia nello schema di Decisione di finanza pubblica? Ancora, il 5 ottobre scorso

un adempimento a cui assolvere scrivendo quattro cifre approssimative, senza alcun reale impegno. Ma se così fosse, questo solenne *iter* procedurale, con annesso ampio dibattito, sarebbe solo una mortificante e umiliante perdita di tempo per il Parlamento! Le chiedo, signor Vice Ministro, di fare chiarezza su questo punto. Le chiedo di dare risposte concrete e di fugare ogni dubbio, anche se dovrà ineluttabilmente scegliere tra due risposte, entrambe scomode per il Governo. Ci sono, infatti, centinaia di migliaia di docenti della scuola e dell'università che non possono accettare risposte contraddittorie ed evasive. Non ci siamo mai rifiutati di combattere gli sprechi, ma questo non vuol dire accettare tagli; nessuna idea: solo tagli che stanno affossando la cultura e la formazione in questo Paese, affossandone anche le prospettive di sviluppo! Del resto, la stessa 7a Commissione, checché ne dica il senatore Valditara,

integrare il fondo per l'offerta formativa, ripristinare le dotazioni del fondo di finanziamento ordinario dell'università, ripristinare gli scatti di anzianità ed estenderli anche all'università.

anche se rinvia, per queste condizioni (in modo ridicolo, perché le condizioni non si fissano per ciò che verrà, ma per ciò che è stato), al disegno di legge sulla stabilità economica. si è costretti a navigare a vista in questo contesto di incertezze, viene approntato uno schema di decreto attuativo dell'articolo 64 della legge n. 133 del 2008, quello sui corsi serali (è importante che i colleghi prendano atto di questo fatto gravissimo) che, se approvato così com'è, rischia di distruggere un'esperienza straordinaria che ha consentito a tanti lavoratori del nostro Paese e a tanti cittadini costretti dalle condizioni economiche a lavorare precocemente di elevare il proprio livello culturale, di inserirsi nel mondo delle professioni, in molti casi frequentando con successo l'università. Siamo dunque disponibili a cercare soluzioni adeguate ma ci troviamo puntualmente solo e soltanto davanti a una logica dei tagli

di questa «indecisione di finanza pubblica» - che questo documento è il primo e l'ultimo del suo genere, allora possiamo dire che esso nasce male e muore ancora peggio. Nasce male perché porta avanti quel processo di svuotamento del ruolo del Parlamento a cui questa maggioranza, e questo Governo, ci hanno già abbondantemente abituato. Lo abbiamo visto con la manovra finanziaria di anticipazione del luglio 2008, presentata come una grande innovazione della politica economica, alla quale hanno poi fatto seguito una miriade di decreti-legge economici che hanno determinato soltanto una frammentazione di presunte risposte. Lo abbiamo visto con il decreto-legge Grecia: quando noi qui in Aula discutevamo dell'aiuto di 5,5 miliardi di euro alla Grecia, il Ministro dell'economia giurava e sacramentava che non ci sarebbero state manovre economiche per il nostro Paese. Ebbene, dopo soli due mesi è arrivata una manovra da 24 miliardi di euro. Lo abbiamo visto poi con l'ultimo decreto-legge, quello del mese di luglio, in cui i tagli alle Regioni e ai Comuni non hanno avuto una condivisione in sede di Conferenza Stato-Regioni. Quindi, a tutto questo noi eravamo già abituati, ma, vede, questo è un documento presentato da una maggioranza che del taglio delle spese, e della spesa pubblica,

lo ricordo a me stesso - prevede espressamente il controllo del Parlamento attraverso l'indicazione di tutte le informazioni utili e necessarie. Ebbene, in questo documento manca l'indicazione delle risorse finanziarie che vengono impegnate per gli interventi e le iniziative nei principali settori di spesa; in questo documento manca il contenuto del Patto di stabilità interna e, cosa ancor più preoccupante in epoca di un federalismo sbandierato e propagandato, manca il patto di convergenza. Questo documento, infatti, non è stato discusso, almeno per quanto riguarda le linee guida, con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, espressamente prevista dalla legge sul federalismo, approvata soltanto un anno fa, per il semplice motivo che questa Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica non è stata ancora istituita. Ma questo documento muore ancora peggio, muore ancora peggio, perché questa crisi economica, che è stata in fondo determinata da una crisi finanziaria provocata dalle grandi speculazioni delle strutture bancarie e delle intermediazioni finanziarie, viene, di fatto, caricata e scaricata sulla pelle dei pensionati e dei dipendenti pubblici. La Decisione La Decisione di finanza pubblica, infatti, dice semplicemente che recepisce tutti gli effetti del decreto-legge n. 78 del 2010. ricordo ai colleghi che il decreto-legge n. 78 prevedeva tagli alla spesa attraverso il blocco delle retribuzioni nel pubblico impiego, attraverso lo slittamento delle pensioni con la chiusura delle finestre, e poi attraverso i tagli alle Regioni, Province e Comuni per un importo di 13 miliardi di euro nel triennio. però che uno dei punti principali della politica economica di questa maggioranza e di questo Governo sia la stabilizzazione dei conti pubblici. anche su questo passaggio ci si deve mettere d'accordo, signora Presidente, signor Vice Ministro, signora relatrice. Bontà vostra, mi dite un solo dato

L'avanzo primario è di segno negativo; il decreto-legge n. 78, per la stessa affermazione del Governo, aveva un effetto recessivo di oltre 0,5 punti in termini percentuali.

quella crescita, produttività e competitività di cui tanto si parla.

Il Governo e la sua maggioranza l'hanno affrontata dimostrando - è una valutazione nei fatti - uno scarso peso politico ed una scarsa autorevolezza a livello degli organismi internazionali. Per mesi siamo stati informati dal Ministro dell'economia che la nuova ridefinizione del Patto di stabilità e crescita europea doveva avvenire necessariamente attraverso l'incontro sul parametro del debito aggregato. È vero che il nostro Paese ha un debito pubblico alto, ma è altrettanto vero - e non per merito di questo Governo - che i risparmi privati sono ancora solidi. Che cosa è stato invece trattato a livello europeo? Il 29 settembre la Commissione europea propone che la rivisitazione del Patto di stabilità e crescita avvenga attraverso una accelerazione del rientro del debito pubblico nei limiti del 60 per cento, accelerazione dell'ordine di un ventesimo per ogni anno. Ciò significa

È bene che gli italiani sappiano che debbono aspettarsi lacrime e sangue, perché saranno varate manovre finanziarie dell'ordine di 30-40 miliardi di euro.

e di razionalizzazione della spesa pubblica, che vengono ancorate agli effetti del tanto decantato federalismo fiscale: signori rappresentanti del Governo, ci troviamo semplicemente ad un decreto e mezzo

andrà probabilmente a regime nel 2014. L'Europa, l'Italia e gli italiani non possono aspettare questi tempi, se non si interviene con altre soluzioni e scelte più coraggiose.

Abbiamo presentato alcune proposte di livello europeo, tra cui - ad esempio - la tassazione sulle transazioni finanziarie, che non è una proposta eversiva, perché è stata fatta dal Governo francese di Sarkozy. Abbiamo presentato la proposta del divieto delle vendite allo scoperto, che non è una proposta eversiva perché è stata avanzata dal Governo tedesco della Merkel. poi le proposte sul fronte interno, come la tassazione sulle rendite finanziarie (esclusi i titoli di Stato), l'aliquota aggiuntiva del 7,5 per cento agli evasori ed elusori che hanno usufruito dello scudo fiscale e tutte

la maggioranza e il Governo abbiano bisogno a questo punto di scelte coraggiose. Non è più il tempo né il luogo per potersi iscrivere al *clan* dei rigoristi, o dei non rigoristi, però non si può andare avanti di rinvio in rinvio, di ritardo in ritardo, di omissione in omissione, perché sta sprofondando il nostro Paese. Mi consenta di concludere, signora Presidente, che, sprofondando una parte signora Presidente, che, sprofondando una parte importante del Paese, noi dell'Italia dei Valori (e credo anche il resto dell'opposizione) consideriamo che a questo punto l'unica capsula Phoenix utile sia rimandare a casa questo Governo.

signori rappresentanti del Governo, il documento di Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 nasce già vecchio e inadeguato. La revisione del Patto di stabilità e crescita su cui sta maturando un consenso a livello europeo rende gli scenari di finanza pubblica prospettati del tutto inadeguati rispetto alle necessità. Si prospetta infatti un aggiustamento più ampio del previsto. Rispetto alle previsioni diffuse dopo il varo della manovra di maggio (e parliamo solo di maggio) emerge già un deterioramento dell'avanzo primario di 0,2 punti del prodotto interno lordo (circa 3 miliardi di euro) per il 2011 e 2012. Ciò è dovuto (cito testualmente dal documento) «a parità di ipotesi di crescita» a una «riduzione del gettito atteso». Insomma, sia le entrate che la crescita vanno peggio di quanto si potesse prevedere nel mese di giugno. Un peggioramento che si è già rimangiato un quarto della correzione effettuata con la manovra e che valeva 0,8 punti di PIL l'anno. È un dato su cui riflettere, soprattutto tenendo conto che la manovra varata in primavera contava sulla possibilità di recuperare più di 8 miliardi per anno dall'evasione fiscale da qui al 2012. Si è addebitata la difficoltà alla crisi internazionale: ma l'unico dato che tira sul versante dell'economia reale è l'andamento dell'*export* e quindi della domanda internazionale. In realtà, l'economia mondiale sta crescendo e parecchio: quella che non cresce è l'economia italiana. Non tira la domanda interna; calano gli investimenti; non c'è una proposta, se non fantasiose ipotesi, per le infrastrutture; non ci sono segnali per far crescere la produttività dei fattori,

tassazione elevatissimo, in aggiunta alla mancanza di una pubblica amministrazione efficiente, ai trasporti inefficienti, a una giustizia civile inesistente. È quanto dice Mediobanca nel suo rapporto dell'altro ieri. Servono riforme strutturali, ma le riforme non ci sono. Serve - lo dico a nome dei componenti del Partito Democratico nella Commissione industria - una politica industriale; ma anche su questo siamo allo zero assoluto, tanto che abbiamo potuto per lungo tempo, in presenza di centinaia di gravi crisi aziendali, con la scomparsa di settori strategici, fare a meno del Ministro dello sviluppo economico. Sviluppo: ecco ciò che non c'è. Non c'è alcuna idea per lo sviluppo. C'è una tecnica comunicativa che, quando la si adotta in qualunque impresa, porta necessariamente prima alla difficoltà e poi al fallimento: si dà la colpa del cattivo andamento all'esterno, si rimandano nel tempo le valutazioni sugli andamenti reali, si spostano in avanti le scelte, non si verificano gli andamenti attuali, come sta avvenendo in questi mesi. E, come sempre accade, gli andamenti attuali non confermano le aspettative. Sul piano sociale, cresce la disoccupazione, crescono le disuguaglianze, cresce l'economia sommersa, cresce la precarietà. Non c'è neppure un segno di emozione per il fatto che un'intera generazione, o forse due, dovranno - come ha detto il governatore Draghi - «saltare il turno». Quello che ci prospettate è un Paese senza euforia, vecchio, patrimonializzato nel suo 10 per cento più ricco, immobile e debole nell'innovazione. Un Paese senza futuro. È un Paese inaccettabile, però, soprattutto per quelle piccole e medie attività economiche, per quel lavoro autonomo che ha scommesso di farcela e non pensava che stare sul mercato volesse dire partecipare ad una fiera nella quale non c'è alcuna regola e nulla di quel sistema che Luigi Einaudi prospettava nelle sue meravigliose lezioni di politica sociale e che raffigurava significativamente nei carabinieri che fanno rispettare le regole, nei vigili urbani che prevengono le liti, nel sindaco e nel segretario comunale che prospettano gli ordinamenti, nella pretura e nella conciliazione che risolvono le diatribe, nelle strade, nelle piazze, cioè nello Stato che, accettando il mercato, non rinuncia a farlo funzionare secondo meccanismi di di concorrenza e di salvaguardia delle regole, cioè non rinuncia ai propri valori. La Decisione di finanza pubblica non contiene indicazioni programmatiche in relazione alle politiche economiche e di settore per i prossimi anni. Si conferma l'impressione che l'azione dell'Esecutivo sia esclusivamente in balia degli eventi e delle contingenze che di volta in volta si manifestano. Al vuoto delle politiche per il sostegno e il rilancio del sistema produttivo si accompagna l'assenza di qualunque politica per lo sviluppo del Mezzogiorno, mentre sono del tutto mancanti opzioni in materia di liberalizzazioni e di tutela della concorrenza e indirizzi per il sostegno e l'attrazione degli investimenti in quei settori quali il turismo, l'*information and communication technology*, le biotecnologie, la chimica fine, le energie rinnovabili - sui quali si dovrebbe puntare per il rilancio della competitività dell'Italia. Noi riteniamo che occorra sostenere e promuovere progetti industriali che guardino al futuro, favorire lo sviluppo dei settori a più alta intensità tecnologica, la *green economy* e la componentistica per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Riteniamo inoltre che occorrano indirizzi e risorse finanziarie per sostenere il turismo,

È necessario ripristinare la piena automaticità delle incentivazioni, quali il credito di imposta per gli investimenti e l'occupazione; bisogna rimettere in campo incentivi per le ristrutturazioni edilizie e per l'efficienza energetica degli edifici. Si tratta stato detto - sostenevano interi settori. Il settore più in crisi nel nostro Paese è quello delle costruzioni: proprio questo settore avrebbe ricavato più vantaggi dalle ristrutturazioni e dall'efficienza energetica. Soprattutto per le piccole imprese permane un'emergenza creditizia. Non è finito, signor Vice Ministro, il *credit crunch* per le piccole imprese; anzi, l'avvento di Basilea 3 fa prevedere la necessità di interventi suppletivi per l'accesso al credito delle piccole imprese, ben più forti di quelli che sono stati messi in campo nella tornata della grande crisi del 2009. Vanno riavviati gli interventi di liberalizzazione dei mercati, per favorire la libera concorrenza concorrenza tra imprese e diminuire i costi a carico del cittadino consumatore (perché non riprendere l'agenda Industria 2015?). Vanno ripristinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, rilanciando il programma degli interventi. cioè rimessa in campo una politica industriale che sia una politica per lo sviluppo e che sia una politica che abbia una visione e dei valori per il Paese. Non va ripetuto costantemente il libro dei sogni che ci viene propinato continuamente e che anche il Presidente del Consiglio in quest'Aula ha di nuovo ribadito. Troppi sogni, ripetuti troppe volte, talvolta diventano degli incubi.

da assumere all'interno del semestre europeo, periodo in cui si darà vita per la prima volta a una sorta di sessione di bilancio comunitaria. La Decisione di finanza pubblica sottolinea come la la crisi economica e finanziaria degli ultimi due anni e la necessità di mantenere gli impegni assunti in sede europea hanno determinato l'anticipazione della manovra di aggiustamento dei conti per gli anni 2011-2013, attuata con la manovra di luglio. Il ministro Tremonti conferma, nella premessa della Decisione di finanza pubblica, che la legge di stabilità sarà «sostanzialmente tabellare e di contenuto assai ristretto». Questo consentirà di evitare di drammatizzare la discussione autunnale sulla finanziaria nell'ambito della sessione di bilancio, superando le prassi complesse e tempestose del passato. Il Ministero dell'economia conferma gli impegni politici definiti con l'Europa e, a tale proposito, puntualizza che l'avviata riforma della politica economica europea fa di questo documento «il primo e l'ultimo del suo genere»: difatti, esso «è (...) sostanzialmente e politicamente superato», visto che i nuovi documenti europei dovranno essere scritti e presentati prima della fine dell'anno e avranno da subito una centralità politica assoluta e assorbente. Va detto che la ripresa che è in atto, più forte in alcuni Paesi come la Germania e più debole in Italia, rischia di non accelerare se non si liberano risorse economiche in grado di rilanciare investimenti investimenti produttivi e sviluppo. Nel complesso, il quadro macroeconomico resta difficile, la ripresa mostra segni di debolezza e restano tensioni sui mercati finanziari, Il controllo della spesa resta cruciale in previsione dell'attuazione del federalismo fiscale, occasione importante per razionalizzare spese e migliorare i servizi resi ai cittadini. È urgente avviare la transizione dalla spesa storica al costo standard; lo è parimenti il rafforzamento della lotta all'evasione fiscale: tutte precondizioni essenziali per avviare la riduzione delle aliquote di imposta per famiglie e imprese, considerato che il prelievo fiscale si conferma nel nostro Paese particolarmente gravoso nel confronto internazionale. Un giudizio positivo va espresso sulle misure volte a rendere più efficiente la pubblica amministrazione e ad elevare l'età di pensionamento per uomini e donne, come è stato rilevato nel corso dell'audizione dal direttore generale della Banca d'Italia. Va detto che la manovra anticipata ha certamente contribuito a dare più certezze agli operatori. Occorre monitorarne gli effetti, in particolare sul fronte della lotta all'evasione. Da questo punto di vista, la stretta sulle compensazioni IVA in vigore dallo scorso 1° gennaio è senz'altro positiva. Quello che si evince dalla Decisione di finanza pubblica è, dunque, una ripresa a ritmo moderato che sconta una permanente stasi dei consumi. L'Italia deve integrare - è stato detto ed occorre ripeterlo - le politiche di rigore con quelle di rilancio dell'economia. auspicabile che, in vista del prossimo avvio del semestre europeo, sia messa a punto una strategia più articolata capace di integrare il controllo dei saldi di bilancio pubblico con iniziative di rilancio delle prospettive di crescita del nostro Paese. Una crescita più lenta acuisce le difficoltà di gestione della finanza pubblica.

«Il Sole 24 ore», che registra in particolare, per quanto riguarda l'occupazione femminile, addirittura una situazione di regresso rispetto ai mesi precedenti. La differenza più rilevante è nella partecipazione alle forze di lavoro, che vede le donne impegnate al 52 per cento, mentre gli uomini raggiungono il 74 per cento. È molto lenta la crescita del peso delle donne sulla forza lavoro complessiva, inoltre un divario particolarmente pesante sopravvive anche a livello di salari, poiché le donne guadagnano in media il 50 per cento degli uomini. La crisi finanziaria, il cui svolgimento è ancora in corso, ha sicuramente insegnato che occorre ridisegnare il mondo delle regole e delle formule finanziarie: non sarà più possibile erogare crediti a pioggia senza una preventiva e ancora più accurata valutazione dei rischi. Il mercato diventerà più selettivo e più rigido. Anche i meccanismi di *rating* dovranno essere ripensati e rimodulati. In questo scenario non si possono dimenticare le nuove regole di Basilea 3, che mirano a rendere più stabile e più trasparente il sistema finanziario nel suo complesso. Tuttavia, i centri di ricerca economica specializzati hanno già calcolato che l'applicazione delle nuove norme stabilite da Basilea 3 potrebbero incidere nel prossimo triennio in ragione dello 0,5-0,7 per cento del PIL europeo. Questo vuol dire che l'applicazione degli accordi non sarà neutrale. Le banche saranno chiamate a rispettare maggiori oneri, che saranno fatti trasferire sulla clientela. Si ridurrà il numero delle piccole e medie imprese che accederanno al credito e il costo dell'ottenimento di capitali Una parte delle risorse finanziarie sarà risucchiata dalla nuova piattaforma di regole, e tutto ciò potrebbe indurre ad un rallentamento della crescita. Diviene, dunque, ancora più importante quanto già anticipato dal ministro Tremonti al *meeting* di Rimini, e quanto va ripetendo, cioè una sorta di decalogo per la crescita, partendo dalla premessa della riforma fiscale; riforma che passa attraverso una drastica semplificazione di regimi e di aliquote da sostenere con interventi concreti diretti alle famiglie, all'impresa, al lavoro e alla ricerca, senza dimenticare il *welfare* e senza dimenticare - lo voglio sottolineare ancora una volta, a proposito di politiche fiscali - tutto ciò che incentiva l'occupazione femminile. L'auspicio è che proprio in previsione della messa a punto dei documenti sui quali si aprirà il confronto europeo a Bruxelles (aggiornamento del programma di stabilità e piano nazionale di riforme) si dia il via in Parlamento a una sessione di confronto costruttivo,

abbiamo sempre detto che la scelta della moneta unica comporta la necessità di mettere in campo altri strumenti di politica economica comune.

gli interessi nazionali, nel nuovo contesto globalizzato, si salvaguardano - appunto - combattendo una battaglia per una comune patria europea. però, il punto è un altro. Infatti, signor Vice Ministro, gli strumenti che l'Europa sta predisponendo per compiere un passo in avanti sono discutibili e rischiano di essere inefficaci, perché hanno il difetto di aggravare la componente prociclica degli

Avete parlato di uno straordinario piano di infrastrutture per il Mezzogiorno: dove sono le risorse se gli investimenti calano nel triennio di più di un punto del PIL,

Ma ciò vuol dire almeno 3 punti di PIL di manovra all'anno; vuol dire avere un avanzo primario di più del 4 per cento; vuol dire tagliare ogni anno tra i 40 e i 50 miliardi di spesa. Ma lo volete dire agli italiani?

Gli statisti fanno così! I politicanti invece hanno paura di dire le cose scomode, che però sono quelle che spesso fanno comodo alla vita degli italiani del futuro.

intervenendo con coraggio, non con quella cosa ridicola del federalismo demaniale, mettendo a risorsa il grande patrimonio pubblico del nostro Paese

Se non cresceremo di più non riusciremo mai ad affrontare il debito che abbiamo sul groppone. Politiche per lo sviluppo. Da noi la spesa pubblica è cresciuta senza interventi di sostegno dell'economia. Certo, è cresciuta anche perché gli ammortizzatori sociali sono stati rifinanziati. Ma perché non avete fatto la riforma degli ammortizzatori sociali? Ci mettiamo dei soldi? Giusto, ma mettiamoceli spendendoli meglio. Crescere di più è un capitolo che non esiste. il segretario generale dell'OCSE, di fronte all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ha illustrato il suo rapporto annuale: ha confermato una crescita incerta si faccia qualcosa per crescere di più. Le parole chiave sono sei: istruzione, ricerca, concorrenza, innovazione, crescita, verde. Cosa c'è nel documento su questi temi? Quello che c'era viene tolto, e di nuovo non c'è nulla. Non avete più fiducia, voi, nel Paese. Ed è il Paese che vi toglierà la fiducia.

Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli senatrici e senatori, la discussione sulla Decisione di finanza pubblica 2011-2013, che da quest'anno sostituisce, e per l'ultimo anno, il Documento di programmazione economico-finanziaria, giunge in una circostanza particolare, ma non per responsabilità del Governo o del Parlamento, bensì per per gli effetti della crisi finanziaria internazionale, che hanno determinato la modifica di tutto il sistema di regolamentazione europea e che, partendo segnatamente dalle condizioni in cui si è trovata la Grecia alcuni mesi or sono, ha portato l'Unione europea a determinare un modello diverso di programmazione che ci porterà al al programma di riforma nazionale fra pochi giorni, con i primi dati che scaturiscono comunque da questa sintetica Decisione di finanza pubblica, e successivamente, di anno in anno, al nuovo programma di stabilità. Questo ha anche determinato, in ambito nazionale, il provvedimento approvato durante l'estate, il decreto-legge n. 78, convertito con la legge n. 122 del luglio scorso, in tal modo i conti pubblici del nostro Paese sono stati posti al riparo da turbolenze ed eventuali iniziative speculative che avrebbero potuto mettere in difficoltà, come è successo appunto

Inoltre, è da rilevare che l'anticipazione delle manovre finanziarie già avviata dal Governo fin dall'insediamento, nel 2008, va incontro a tutte le tendenze già emerse a livello europeo. Quindi la nuova periodizzazione periodizzazione che si avrà a livello europeo serve proprio a creare le condizioni per determinare in modo poi tempestivo e uniforme a livello europeo gli indirizzi di governo dell'economia. Nondimeno, l'attuale documento costituisce una rilevante opportunità per puntualizzare le azioni condotte dal Governo per contrastare la crisi finanziaria internazionale e per garantire la sicurezza dei conti pubblici, in relazione all'evoluzione dell'economia italiana. Quest'ultima è, in realtà, il vero oggetto su cui puntare l'attenzione, nella consapevolezza che l'azione dei pubblici poteri può sì stimolare un *trend* di crescita e parzialmente indirizzarne l'evoluzione, ma l'elemento di base è rappresentato dalla capacità di reazione del sistema produttivo ed economico rispetto alle sfide che vengono lanciate dal mercato. Oggi, la domanda che non solo gli economisti e i politici si pongono, ma anche i cittadini, è se la peggior crisi finanziaria da settant'anni a questa parte sia passata o se siano ancora concreti i rischi di una ricaduta secondo il modello a "W", com'è stato definito da taluni esperti. È indubbio che il culmine della crisi sia stato superato e che ora si tratti di affrontare le conseguenze di questo evento, ponendo le basi per un recupero quanto più veloce possibile ma, soprattutto, fondato su basi solide, tali da evitare che i meccanismi di speculazione finanziaria possano possano ancora minare, in un futuro non lontano, i fondamenti dell'economia reale. In primo luogo, occorre che sia definito, a livello internazionale o quanto meno europeo, un piano di smaltimento graduale dei debiti pubblici accumulatisi per far fronte alla crisi. Vorrei ricordare che la gran parte dei Paesi d'Europa (non l'Italia, perché non poteva; non l'Italia, perché

A loro volta, le entrate dello Stato sono naturalmente influenzate dall'andamento dell'economia, in un gioco intrecciato che richiede attenzione e prontezza d'intervento. Il conto economico delle amministrazioni pubbliche - come bene ha esposto la relatrice, senatrice

Complessivamente, nel primo semestre del 2010 si è registrato un indebitamento netto pari al 6,1 per cento del prodotto interno lordo, in riduzione rispetto al valore del 6,3 registrato nel primo semestre del 2009. Sempre nel primo semestre, il saldo primario rispetto al prodotto interno lordo, cioè al netto degli interessi passivi, è negativo e pari all'1,5 per cento, valore identico a quello registrato nello stesso periodo dell'anno precedente; naturalmente, questo è negativo, ma va valutato nel contesto mondiale. Sempre nel primo semestre del 2010, le entrate totali risultano diminuite dello 0,8 per cento, mentre si erano ridotte

il livello di imposizione fiscale complessivo rispetto al prodotto interno lordo, e non solo enfatizzare in negativo quando sale. Si denota dunque un andamento migliorato, per effetto incrociato del recupero dell'economia italiana con i provvedimenti messi in atto dal Governo, sia di stimolo verso taluni settori, sia di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Nel complesso, si è rilevata una tendenza espansiva dell'economia abbastanza sostenuta per la metà dell'anno, per poi assistere certamente a una fase più riflessiva e contenuta nel terzo trimestre. Altrettanto positive considerazioni si possono fare analizzando i dati relativi al fatturato e agli ordinativi dell'industria nel confronto degli ultimi tre mesi con i tre mesi immediatamente precedenti

L'indice del fatturato, in particolare, ha registrato a luglio un incremento dell'8,9 per cento rispetto all'anno precedente. Naturalmente si rileva che il recupero è ancora parziale rispetto ai livelli produttivi ante crisi. Nel confronto tendenziale relativo al periodo gennaio-luglio, l'indice del fatturato ha segnato un aumento dell'8,1 per cento, confermando quindi tutte le preoccupazioni circa la velocità di una ripresa che non appare ancora completamente consolidata; altrettanto si può dire per il settore dei servizi. Di fatto, nel dettaglio delle attività economiche si coglie la rilevanza che finora ha avuto l'*export* per stimolare gli indici positivi fatti registrare nell'anno; si parla del 12-12,5 per cento di incremento e questo è il primo dato sostanziale. Certamente bisogna anche ricordare, dall'altra parte, che all'aumento delle esportazioni corrisponde anche un aumento delle importazioni e, quindi, di un deficit, ma questo è un dato positivo perché, essendo l'Italia un Paese trasformatore, è automatico che la ripresa è accompagnata nell'immediato dall'aumento delle importazioni. Un andamento stagnante - bisogna ricordare - si ha ancora sui consumi interni, che costituiscono al momento attuale l'elemento di freno; ma ciò accade non solo in Italia, ma in tutta l'Europa. La giustificazione di tali comportamenti di consumo è facilmente rinvenibile nel quadro ancora instabile dell'occupazione, quale si è fermata sul livello della disoccupazione ma purtroppo fa crescere anche i soggetti inattivi. Signora Presidente, concludendo, in questo quadro si può rilevare come ci sia un equilibrio che passa attraverso la riduzione della pressione fiscale e che dà sicurezza: azioni graduali, ma ferme. Non si può nascondere, però, il ruolo, decisivo a mio avviso, che dovrà avere, per la ripresa economica, la capacità del Paese nel suo complesso di imboccare una direzione di crescita a ritmi più sostenuti

il nuovo documento relativo al quadro degli obiettivi e delle previsioni economiche di finanza pubblica fornisce qualche osservazione sulle principali questioni emerse nel corso del dibattito. A partire da quelle più «politiche», come ad esempio le motivazioni per le quali il documento non contiene alcune informazioni previste dalla legge di contabilità, ritenendosi che le possibili carenze informative siano individuabili soltanto nelle novità procedurali e contenutistiche dei documenti stessi, che, probabilmente, si riflettono anche a livello delle amministrazioni coinvolte nella indicazione delle stesse. Mi sembra più rilevante, invece, prendere in considerazione l'affermazione del Governo nella sua relazione di accompagnamento circa il superamento sostanziale del documento in esame.

mi permetto di correggerla: mai nessuno ha definito questo documento irrilevante. Certo, per stessa indicazione del Governo, è un documento che mostra il suo superamento dal punto di vista politico, ma non economico. Questo ritengo non debba leggersi come un volerne sminuire il significato (che gli è stato conferito da una legge), ma solo come un voler prendere atto del fatto che questa prima applicazione della riforma contabile si trova nel mezzo di una manovra già attuata e delle profonde innovazioni alla *governance* economica comunitaria che si vanno definendo in sede europea. Della quale ricordo che è in corso la fase transitoria, in cui sono previsti incontri bilaterali con la Commissione europea per approfondire gli aspetti procedurali e contenutistici del piano nazionale di riforma.

oggetto invece di ulteriori e necessari approfondimenti da condividere in sede Europa, e non solo da parte del Governo. Tra l'altro, vorrei ricordare al senatore D'Alia che la nuova legge di contabilità non è mai stata da noi considerata la panacea di tutti i mali: avremmo peccato di un eccesso di illuminismo! Si è trattato invece convintamente della necessaria riforma di una normativa complessa e farraginosa, che non abbiamo esitato, tutti, a criticare nel corso di questi ultimi anni. Per quanto riguarda i contenuti, dico subito che il vero punto debole di questo documento è costituito dal dato relativo alla spesa per investimenti, che è in diminuzione: una tendenza che a mio avviso va necessariamente e rapidamente invertita. Siamo perfettamente consapevoli che non può esserci ripresa senza adeguati investimenti, soprattutto nelle infrastrutture, quelle materiali e quelle immateriali, anche nella precondizione dell'attuazione del federalismo fiscale, di quel riequilibrio territoriale necessario che ci ha ricordato il senatore Fleres. Resto convinta che il completamente e l'accelerazione dei tempi di realizzazione della TAV siano strategici e fondamentali per trattenere la potenzialità del corridoio 5 al di sotto delle Alpi, ma che sia lei, senatore Marco Filippi, a bacchettarci sui ritardi accumulati mi fa proprio specie! Posso ricordarle senza tema di smentita la scellerata attività svolta dal ministro dei lavori pubblici Di Pietro di quel Governo Prodi, che lei sosteneva con tanta passione, che in cinque minuti cancellò il lavoro di cinque anni.

n. 78, che garantisce il finanziamento incrociato per le opere ferroviarie connesse al potenziamento della tratta Verona-Fortezza, porta strategica del traforo del Brennero, l'opera più rilevante, dal punto di vista

Il conseguimento possibile del 5 per cento del disavanzo nel 2010 costituisce, infatti, un vincolo imprescindibile. Il riequilibrio del bilancio viene per noi prima di tutto; la tenuta dei conti pubblici è il presupposto senza il quale ogni altro provvedimento volto a sostenere la crescita perderebbe di efficacia. Pensi, senatore Mascitelli se non avessimo fatto quei tagli che tanto ci avete criticato proprio per tenere in ordine quei conti pubblici, oggi cosa ci troveremmo ad affrontare. E, senatore Mercatali, non abbiamo mai creduto che i tagli fossero l'unica medicina, ma di certo il presupposto per riqualificare e migliorare la spesa pubblica. È il mercato purtroppo, senatore Mascitelli, che ha stabilito che la manovra economica del Governo italiano in questi ultimi anni è stata tra le più efficaci d'Europa, che il *rating* di tutti i Paesi è stato abbassato e svalutato ad eccezione del nostro. Ci sarà un motivo se i mercati ed il *rating* apprezzano questa scelta e non ci penalizzano nelle fasi delicate, quelle che espongono altri Paesi a a dissennate speculazioni. Vorrei augurare anche a lei, senatore Mascitelli, che questo Governo non andasse a casa. Guai se questo Governo smettesse la sua azione, non solo riformatrice ma di grande contenimento e di assunzione di responsabilità, così come ha fatto finora! I dati li abbiamo illustrati ieri a proposito di quella pressione fiscale che è uno dei temi qualificanti della nostra azione. Vorrei far presente che ci stiamo riavvicinando a quel 42 per cento

con una non condivisibile politica basata, come al solito, sull'incremento della spesa pubblica. Ricordo solo le tanto vituperate stabilizzazioni, che sono costate decine e decine di milioni di euro ai contribuenti italiani quando lei, senatore Cabras, sosteneva il Governo Prodi tutto basato sulla filosofia del *tax and spending*. Certamente, non penso che non si possa e non si debba fare meglio. Per incidere significativamente sulla pressione fiscale complessiva occorre secondo noi mettere mano alla non più rinviabile semplificazione e ammodernamento del nostro sistema tributario, traducendo in realtà la filosofia espressa dal ministro Tremonti dello spostamento del carico fiscale dalle persone alle cose: una vera e propria rivoluzione, obiettivo irrinunciabile del nostro Governo. Una filosofia che consentirà di superare le criticità operative che pone la capacità contributiva: concetto ovvio, come si è evidenziato nel tempo, però sempre difficile da definire oggettivamente. Spostare il tiro verso il prelievo sulle imposte indirette rende più stretto il nesso tra manifestazione della ricchezza e la sua dovuta tassazione. L'obiettivo, come ricordavo nella relazione relazione di apertura dei nostri lavori, è la riduzione delle tasse, che necessita di azioni di sistema per essere conseguita al termine di un percorso di semplificazione e di disboscamento dell'intricata palude del nostro sistema tributario, che ha come sede di piena valorizzazione il percorso del federalismo fiscale, anche se qualche risultato, a mio avviso, potrebbe essere conseguito fin da subito: ad esempio, esonerando dal pagamento dell'IRAP le micro imprese. Le risorse così recuperate potranno poi essere ulteriormente integrate da quelle derivanti da un contrasto effettivo e puntuale all'evasione fiscale, un'attività che questo Governo ha già intrapreso, con risultati che ad oggi sono certamente lusinghieri. Certo, la situazione della nostra economia migliorerebbe nettamente, con meno evasione e con meno sommerso, ma siamo anche consapevoli di un fatto. Nonostante gli ultimi dati delle Agenzie delle entrate, particolarmente incoraggianti, evasione e sommerso dipendono anche da regolamentazioni esasperanti, da pesi fiscali eccessivi e dalla sensazione che una parte di ciò che viene conferito al fisco sia spesa molto male. La crescita del nostro sistema passa attraverso un incremento della domanda, che può avvenire innalzando il reddito a disposizione di persone e famiglie ma non con alchimie e sostegni di breve respiro, bensì attraverso una politica basata non solo sulla riduzione del carico fiscale - attraverso quel quoziente familiare che vogliamo perseguire con grande forza, senatore Barbolini - ma anche attraverso il rafforzamento delle retribuzioni. Un obiettivo che, per il settore privato, passa certamente da nuove e più confacenti relazioni industriali e nuovi modelli di contrattazione, che diventano strategici per la difesa e l'incremento dei posti di lavoro. Consapevoli però che questo Governo può intervenire con misure di accompagnamento, ma che il ruolo decisivo spetta al mercato e, soprattutto, alle parti sociali. Infatti, sono in corso tentativi tra le parti sociali di definire nuovi assetti del rapporto tra impresa e lavoratori. Penso alla definizione tra le parti sociali di un modello possibile di partecipazione dei lavoratori agli utili, che attendiamo con molta attenzione. Penso al cosiddetto modello Pomigliano, che può dare una risposta concreta alla produttività del lavoro, tema che ci ha ricordato il senatore Morando, ed alla competitività del sistema industriale. A patto, però, che nessuno indugi in atteggiamenti equivoci di complicità con chi, invece, sulla vicenda di Pomigliano cerca ancora di salvaguardare un vecchio armamentario ideologico ampiamente sconfitto dalla storia, dal mercato e dalla parte più coraggiosa e riformista del sindacato italiano. Nessuno pensa di far lavorare le persone come in Cina, ma piuttosto come in Germania: quella Germania che molti evocano a corrente alternata, quando fa comodo e quando no. Alle preoccupazioni cariche di *pathos* espresse dal senatore Treu, che ho ascolato con attenzione (del quale ricordiamo la prima vera grande riforma del mercato del lavoro, con l'istituzione di contratti atipici come i co.co.co.) rispondo con l'invito a guardare la straordinaria positività dei dati italiani sulla disoccupazione rispetto a quelli internazionali, che non solo evidenziano il dato migliore in assoluto del tendenziale italiano, ma che dimostrano persino l'inversione di tendenza che vede diminuire (anche se di poco) la disoccupazione, come primo piccolo segnale di una ripresa economica che si comincia ad intravedere. Lei che è abituato a guardare a fondo i dati, senatore Treu, non può non accompagnare la lettura del dato sulla disoccupazione giovanile giovanile con le modificazioni sociali intervenute nel segmento dai 15 ai 24 anni. Non da ultimo, l'obbligo scolastico (ed io aggiungo per fortuna). Del resto, i bamboccioni non li ho inventati io, ma il Ministro dell'economia del Governo Prodi, che anche lei sosteneva e che portò attenzione la grande responsabilità che avevamo nel consentire ai nostri giovani di allungare a dismisura i tempi, ad esempio, del conseguimento della laurea.

chi avvia un percorso di studio debba completare la sua formazione per accelerare i tempi di ingresso nel mercato del lavoro. Però, prima di far pagare agli studenti quell'eccesso di costo che, invece, oggi è a carico dello Stato nell'allungamento dei tempi, noi abbiamo preferito giudicare con un po' più di severità quei professori e tutto quel corpo accademico, che in saputo solo appesantire il nostro sistema universitario a danno innanzitutto dei nostri studenti.

quanto ricordato dal ministro Gelmini in quest'Aula non più tardi di una settimana fa. Per brevità di tempo non citerò al senatore Procacci il contenuto ed il testo del comma 9 dell'articolo 64 della famosa manovra del 2008, la prima grande manovra economica di questo Governo,

nonostante le indicazioni della tabella di questa Decisione di finanza pubblica, anche la volontà del Governo e del Parlamento, di mantenere l'impegno assunto, che porta a coprire quel mancato blocco con i risparmi conseguiti grazie al contenimento delle spese per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola. E, in riferimento alle donne, signora Presidente, accolgo volentieri una segnalazione contenuta nell'intervento della senatrice Blazina. Non sarò certo io a sottrarmi ad un giudizio critico sull'inefficacia di vecchie politiche occupazionali che mai sono riuscite ad accompagnare le donne di questo Paese verso una maggiore partecipazione al mercato del lavoro. Non so se sia più utile citare i dati dello studio di Goldman Sachs, ma voglio fare ancora riferimento alla ricca elaborazione di tante donne della sinistra storica e di quella sociale che

una donna che per prima arriva ai vertici della vigilanza del nostro sistema del credito - che ricordo essere uno dei più importanti al mondo - qual è la responsabile della vigilanza della Banca d'Italia, Anna Maria Tarantola, proprio ieri ci ha ricordato dalle pagine del «Corriere della Sera»

ma stiamo facendo un favore al Paese che non può più permettersi di avere il 50 per cento di talenti femminili inutilizzati».

quando da questo Governo, come da qualsiasi altro, io attendo la presa di coscienza di questo importante giacimento di capitale umano per conquistare più crescita, più coesione sociale in quella modernizzazione che è la vera cifra delle riforme già fatte e di quelle ancora da fare, ma nell'ottica di una modernizzazione che passerà inevitabilmente, inesorabilmente, in ogni comparto della nostra vita sociale, pubblica e privata, dalle donne di questo Paese.

che si trova immerso in una crisi drammatica e paga un prezzo più pesante di altri alla grande recessione

molto bassa - il dibattito che abbiamo sviluppato in questi due giorni costituisce la conferma più esplicita della profondità della crisi politica nella quale versa il Governo e la maggioranza, soprattutto a causa del venir meno della funzione di guida del Popolo della Libertà, ossia il partito asse del centrodestra, con la drammatica frattura interna e soprattutto a causa di una evidente crisi di *leadership* del leader del centrodestra, cioè del Presidente del Consiglio.

12 novembre, tra meno di un mese, il Governo dovrà presentare in Europa la versione preliminare del Piano nazionale di riforma:

Noi vi abbiamo chiesto di utilizzare l'occasione del dibattito sulla Decisione di finanza pubblica esattamente per avviare questo confronto. Quali riforme verranno proposte tra meno di un mese dal Governo italiano all'Europa, nel contesto della nuova sessione di bilancio europea volta al coordinamento delle politiche economiche e fiscali, che è la

e contiene a tal proposito, signora Presidente, un accenno che immagino sia di involontaria ironia. Si dice, infatti, ad un certo punto della risoluzione della maggioranza l'attuazione del "semestre europeo" dovrà prevedere un tempestivo coinvolgimento del Parlamento nelle diverse fasi di formazione dei documenti da presentare in sede europea, È una settimana che qui al Senato ci sforziamo di dirvi che effettivamente esiste un problema di coinvolgimento tempestivo del Parlamento nel confronto sulle decisioni da presentare in sede europea. Volete approfittare della Decisione di finanza pubblica per iniziare questo confronto? La risposta è stata negativa e - colleghi della maggioranza, signor Vice Ministro, lo capisco - non per cattiva volontà. È la manifestazione classica di una impotenza: voi non potete discutere delle riforme da realizzare nei prossimi mesi ed anni in Italia perché avete perso

nella quale, per due anni, avete detto che durante le crisi non si fanno riforme. Adesso che la crisi si sta un po' allontanando, comincia ad essere alle nostre spalle, pensate di ovviare alla vostra debolezza politica utilizzando la costruzione di un nuovo vincolo europeo. Se guardiamo al passato recente del Paese, vediamo che, per debolezza della politica italiana (di centrodestra e di centrosinistra) ci siamo dimostrati capaci di capaci di produrre cambiamento e di guidare il Paese alla realizzazione di un processo di cambiamento quando abbiamo utilizzato il vincolo europeo. In particolare esso è stato utilizzato positivamente dal primo Governo Prodi in quella fase (1996-1998) che ha salvato l'Italia dall'emarginazione nel contesto europeo. Ma la debolezza della politica italiana è stata tale per cui, appena venuto meno quel vincolo, abbiamo intrapreso immediatamente sentieri divaganti rispetto al progetto di cambiamento di cui il Paese ha Paese ha bisogno e che poi nelle consultazioni elettorali (naturalmente ispirate da valori tra loro alternativi e da interessi sociali anche diversi) sia il centrodestra che il centrosinistra presentano al Paese. La ragione del distacco progressivo

non abbiamo la forza di fare nulla, ma ci sarà l'Europa che ci imporrà delle scelte. A quel punto, grazie al vincolo europeo potremo presentarci in Italia e cambiare qualcosa, fare qualcosa per sollevare il Paese dalla situazione di difficoltà. Ora, per intenderci, questo disegno

Siamo il secondo Paese manifatturiero d'Europa e siamo uno dei più importanti competitori nel campo della produzione manifatturiera nel mondo. Il primo Paese manifatturiero d'Europa e il principale, in rapporto alla sua ricchezza nazionale, Paese manifatturiero del mondo è la Germania. Se ci muoviamo nel contesto europeo semplicemente per subire le decisioni orientate dal gigante tedesco, è probabile che possiamo ricavarne qualche utile in termini di stabilizzazione del nostro sistema finanziario, ma siamo certi che subendo soltanto gli orientamenti della Germania

vedere ridotte le potenzialità di competizione del loro grande competitore in Europa nel settore manifatturiero obiettivamente ce l'hanno, e sarà difficile che resistano a questa tentazione, se sarà loro dato di avere di fronte un interlocutore debole.

volto ad individuare le riforme strategiche necessarie per impedire il declino del Paese e per avviarlo su di un sentiero di stabile crescita. Noi sotto questo profilo abbiamo fatto lo sforzo di presentarvi un disegno: terapia *shock* sul debito pubblico, riforme strutturali dei mercati, equilibrio tra questi due interventi in un disegno di ripresa e di sviluppo del Paese.

finanze*. Signora Presidente, onorevoli senatori, voglio anzitutto ringraziare i numerosi intervenuti a questo dibattito, nel quale, in realtà, delle critiche e dei rilievi che concernono due fattori principali: una presunta inerzia del Governo e una dichiarata mancanza di coraggio. per coraggio: dare corso a spese senza copertura finanziaria (cosa che vorrei scongiurare)? E l'inerzia cos'è? Non fare quello che altri chiedono? Non è così.

lo sviluppo si ottiene con la spesa pubblica, oppure con un solido sistema di finanza pubblica e tenendo sotto controllo gli andamenti della spesa pubblica? Se sviluppo significa maggiore spesa (ad avviso di alcuni), questa poi non finirebbe per riflettersi in un aumento della spesa corrente sotto la voce dell'incremento della spesa per interessi per far fronte alle maggiori spese? La solida finanza

La spesa pubblica aumentata oggi in realtà non è altro che un incremento

vuole cercare anzi di rimediare ai danni che sono stati fatti in passato alle nuove generazioni, ritornando in qualche modo ad una sana e corretta gestione della cosa pubblica,

In realtà, signora Presidente, se vogliamo ben vedere quello che è accaduto negli ultimi due anni, forse non saranno state fatte tutte le riforme desiderabili, però se se non altro sono state realizzate quelle che potremmo definire le madri di tutte le riforme. Mi riferisco segnatamente a due riforme: il federalismo fiscale e la riforma dei bilanci pubblici. Il federalismo fiscale non solo darà una nuova struttura al complesso della pubblica amministrazione italiana (anche per quanto riguarda il lato finanziario), ma consentirà soprattutto di passare ad una diversa impostazione, da quella relativa al costo storico (quindi una sorta di bilancio che tralaticiamente si riportava di anno in anno, creando delle

di diminuire le spese e di razionalizzare i servizi, offrendo dei servizi migliori ai nostri cittadini. Si tratta di due obiettivi che si cerca di conseguire con uno strumento unico, che sarà fondamentale per un rinnovamento complessivo della pubblica amministrazione.

introducendo norme più rigorose per quanto riguarda la copertura finanziaria delle leggi; in sostanza, essa ha la funzione di far cessare quell'assalto alla diligenza che troppo spesso abbiamo visto in passato e che troppo spesso ha creato dei problemi che ancora ci portiamo avanti nelle finanze pubbliche. la nuova legge di contabilità ha consentito di staccare la spina dal bancomat della spesa pubblica, che ci ha portato all'esplosione di un debito con il quale oggi dobbiamo confrontarci la legge di stabilità per il 2011 e per gli anni successivi che sarà approvata oggi dal Consiglio dei ministri va in questa direzione. non manca il coraggio semplicemente per il fatto che dobbiamo tenere dritta la barra della spesa pubblica. Occorre domandarsi se il coraggio sia quello

Certamente l'epoca è difficile e le decisioni da prendere non sono popolari, ma credo che se non si assumono decisioni impopolari, il Paese avrà poche possibilità di sviluppi seri in futuro.

all'andamento della produzione industriale e quelli relativi all'occupazione, preoccupazioni ce ne sono, ma si tratta di dati che, tutto sommato, nell'attuale temperie possono indurci a un certo ragionevole ottimismo anche per il futuro.

alquanto positivo del gettito IVA, a riprova che i consumi interni si stanno riprendendo e che dunque l'economia sta girando in modo ragionevole. Molti hanno lamentato una presunta carenza della lotta all'evasione fiscale. Se guardiamo invece ai dati relativi a una lotta all'evasione - magari fatta

probabilmente più equo, che consente anche di diminuire la pressione fiscale, in prospettiva, nei confronti di tutti gli altri contribuenti. nella gestione di una politica economica come la nostra non esistono né bacchette magiche né scorciatoie, ma bisogna cercare di lavorare al margine, il che comporta minori effetti roboanti, ma più solidi approcci finanziari.

mantenuto nel bilancio a legislazione vigente che sarà presentato nei prossimi giorni al Parlamento, bisogna riuscire a seguire la stella polare per la guida di tutti i conti pubblici, affinché la

affinché una pressione fiscale diminuita possa determinare, tramite un meccanismo di incentivo al risparmio, all'investimento e al consumo, lo sviluppo del Paese con una cifra percentuale superiore a

da un approccio culturale che ormai è giunta l'ora di superare, anche con riferimento alla gestione della finanza pubblica. I Parlamenti sono nati proprio per limitare il potere del sovrano nel richiedere le tasse: dopo aver trascorso anni, decenni e forse anche secoli a fare esattamente l'opposto, cioè a cercare di aumentare la spesa pubblica, potrebbero giustificare il loro permanente valore proprio nel ritorno alle origini,

di avvicinare il momento della Decisione di finanza pubblica a quello della legge di stabilità, per evitare che - come accadeva in passato - tale Decisione venisse assunta molti aspetti dei fenomeni economici che si verificavano durante l'anno, e poi postulava - come tutti i senatori ricordano - la necessità di una nuova sorta di minidecisione a ridosso della vecchia legge finanziaria. Si è pensato, pertanto, di avvicinare i due momenti. invece, ha ritenuto, anche per far fronte alla crisi, di modificare il proprio approccio e passare da una vigilanza *ex post*, sulla base dei risultati dell'economia dei singoli Paesi (quando cioè ormai non c'era più nulla da fare, se non intervenire con un'attitudine sanzionatoria), ad una vigilanza *ex ante*, per evitare

molto difficile essere incoerenti con noi stessi, nel momento in cui coordiniamo le nostre politiche con quelle europee. malgrado le difficoltà esistenti e le molte critiche avanzate, l'Europa sia ancora un continente vivo, in grado di offrire una reazione forte in un momento di difficoltà nel quale bisogna manifestare la propria presenza. E questa reazione europea,

facciamo una prima operazione che chiamerei di tipo einaudiano, cioè diciamo al Governo di fare questa azione di riduzione a partire dall'esigenza di gravare meno sui produttori e un po' di più su altre basi imponibili che poco hanno a che fare con la crescita e la produzione. Quindi, oltre a diminuire la pressione fiscale, invitiamo a redistribuirla tra le diverse basi imponibili, favorendo il lavoro.

aiutiamo il Governo, nel senso che lo rendiamo più forte con un atto di indirizzo parlamentare. Si chiede di utilizzare tutte le risorse provenienti dal successo nella lotta all'evasione fiscale per ridurre la pressione fiscale sui contribuenti leali, evitando che l'aumento di gettito sia usato per finanziare nuova spesa pubblica. Mi aspetto francamente un parere favorevole, sia da parte del relatore sia da parte del rappresentante del

l'emendamento 5.7 proponiamo che nella vostra proposta di risoluzione si espliciti un intervento a favore delle famiglie più numerose e si accetti l'impostazione della richiesta di *no tax area* avanzata di recente dal *Forum* delle associazioni familiari. Sappiamo che c'è uno squilibrio forte nel sistema fiscale italiano tra chi paga e chi non paga, tra lavoro, impresa, grandi rendite e grandi patrimoni, e tra chi ha famiglia e chi non ce l'ha. La famiglia è un valore della convivenza civile, è il primo presidio della coesione e della solidarietà sociale. Il *Forum* delle associazioni familiari ha riconosciuto che il sistema del quoziente familiare costa troppo ed è squilibrato dal punto di vista redistributivo. Si è dunque mosso su una strada molto interessante, vicina anche alla proposta che facciamo di un sistema di interventi fiscali basato sulla cosiddetta dote familiare e sul riconoscimento del valore del lavoro femminile, soprattutto delle donne con figli, con un abbassamento figli, con un abbassamento della prima aliquota. Avete detto che volete fare un piano per la vita e per le famiglie. Accettate questo emendamento, che almeno dà qualche seguito alle promesse che avete fatto al Paese.

del credito d'imposta per le imprese che sostengono dei costi per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo; per i datori di lavoro che incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese; per i datori di lavoro che incrementano il numero di lavoratori e lavoratrici dipendenti di età inferiore ai 30 anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato; di lavoro a tempo indeterminato; per le imprese agricole ed agroalimentari che effettuano investimenti di promozione pubblicitaria in mercati esteri (naturalmente il riferimento normativo che indichiamo è quello della legge n.

il consueto emendamento perché anche le imprese agricole debitrici che non hanno provveduto a richiedere il codice CAR possano provvedere entro il 30 marzo 2011, versando l'importo alle società con modalità regolarmente indicate. È un emendamento che nei contenuti si conosce bene ma che non so per quale motivo non si riesce mai a far andare avanti.

sono strettamente ancorate all'abbattimento del nostro debito, più volte citato come il vero nostro grande punto di debolezza. E alla certezza della redistribuzione del carico fiscale non corrisponde una medesima certezza delle maggiori entrate dovute alla lotta all'evasione fiscale. Ad ogni buon conto, comprendendo lo spirito di questo emendamento, rimetto al Governo la valutazione che vorrà indicare

se incentivate a tal fine. Ritengo che tutto questo vada accompagnato all'interno di un quadro più complessivo di riforma fiscale

nel corso della cosiddetta prima Repubblica, moltissimi provvedimenti erano coperti con i presunti proventi della lotta all'evasione: il risultato è stato che la spesa si faceva, ma le entrate non arrivavano.

revisione complessiva del sistema fiscale, che dovrà tener conto, per essere attivata, dell'andamento della spesa pubblica, e non necessariamente deve essere quella coincidente con il *forum* delle associazioni.

di tutte le parti politiche che in qualche modo hanno appoggiato la Decisione di finanza pubblica - non scende così nel dettaglio, come non lo fa in molti argomenti simili o anche di importanza pari o analoga.

tenere ferma la barra della finanza pubblica, diminuire la spesa e poi fare in modo che le risorse disponibili siano utilizzate a fini di sviluppo. Definire già in questa sede indicazioni di spesa

provvedimenti che ad essa seguiranno. Credo sia più opportuno lasciare alla discussione di quei provvedimenti la definizione delle misure concrete che dovranno immancabilmente essere adottate anche per lo sviluppo del Mezzogiorno, insieme allo sviluppo complessivo del Paese.

Abbiamo sentito che il Governo non intende provvedere in alcun modo alla riduzione del carico fiscale, né per le imprese né per le famiglie.

è che il Governo venga in Aula senza alcuna possibilità di discutere e di trattare il merito dei provvedimenti. Il Governo dice sempre di no. Noi proponiamo qui un'elementare misura, cioè che il ricavato della lotta all'evasione vada alle famiglie e alle imprese: mi sembra che lei non abbia dato alcun elemento di fatto per sostenere l'impossibilità di tale misura. Chiedo alla Presidenza del Senato Senatore Zanda, essendo questa una dichiarazione di voto, ne deduco che insiste per la votazione

Molti dei problemi del Paese si risolvono intervenendo anche sulla domanda interna. Occorre un intervento a favore delle famiglie più deboli, e questa è una proposta molto concreta. Prendiamo atto che anche questo ennesimo nostro tentativo si ridurrà in un fallimento, perché da parte vostra non c'è alcuna disponibilità ad andare incontro alle famiglie, anche quelle che hanno redditi bassi e un carico familiare molto rilevante.

per confondere le idee. Ed avendole confuse persino a lei, immagino quanto riescano a confonderle agli altri. Non ho nulla a che vedere con un Gruppo che è un'invenzione di questo Governo.

al credito d'imposta, così come sento dire dalle imprese del Mezzogiorno d'Italia, immagino che anche i miei colleghi del PdL, che spesso trovo agli incontri con le piccole e medie imprese del Mezzogiorno, abbiano promesso la stessa cosa che ho promesso io. Io l'ho tradotta in emendamento. Se si vuole che le promesse diventino dei fatti, mi auguro che si possa votare in maniera libera, liberi da vincolo di mandato, un emendamento del del cui contenuto si parla spesso e per il quale si assumono anche impegni in più occasioni ufficiali. non c'è nessun riferimento a quel piano per il Sud che pure era stato enunciato sia alla Fiera del Levante dal ministro per gli affari regionali Fitto, sia qui in Aula dallo stesso Presidente del Consiglio. Se almeno si volesse intervenire su una cosa sola che possa minimamente alleviare le imprese del Sud credo che, in fin dei conti, non sarebbe un grande sforzo da parte di questo Governo.

comprendo pienamente e condivido le ragioni della collega Poli Bortone. Mi permetto di ricordare che il credito d'imposta, signora signor Vice Ministro, è stato operante in Italia sino al 2001. Mi permetto altresì di ricordare che quelli sono stati gli anni in cui gli anni in cui il PIL delle Regioni meridionali è cresciuto più che nella media del Paese: vuol dire che sono stati anni in cui vi è stata, obiettivamente, una riduzione del *gap* tra il resto del Paese ed il Mezzogiorno. Si tratta di un incentivo automatico non soggetto ad alcun controllo, né di tipo politico, né di tipo burocratico (e lei, Vice Ministro, sa perfettamente cosa vuol dire questo, in particolare nel Sud del Paese). Paese). È un incentivo che premia le aziende che producono ricchezza: non quelle che investono, ma quelle che fanno un investimento che produce ricchezza.

Signora Presidente, vorrei sostenere anch'io la bontà della proposta della senatrice Poli Bortone, e non solo perché vi è un rapporto sempre più stretto tra il Movimento Io Sud e il Movimento per le Autonomie, ma perché la vicenda del credito di imposta è assolutamente dubbi sulla giustezza dello strumento. È uno dei pochi strumenti, come ricordava bene anche il collega Bianco, che ha dato risultati significativi nell'innescare processi di sviluppo virtuosi, anche in ragione del suo automatismo, ed è stato oggetto, da parte del Governo, di una disattenzione che ha determinato il venir meno del finanziamento per la parte relativa agli investimenti e all'occupazione.

non mi sottraggo a un rapporto dialettico e critico rispetto alla disattenzione che il Governo ha per il Mezzogiorno, attestata dal fatto che, pur avendo affermato, in varie occasioni, all'interno di questo

si sta costruendo una fiscalità di vantaggio al contrario. Come sanno gli amici della Lega Nord con i quali abbiamo conversato, immaginare di autorizzare le Regioni con i conti in ordine ad azzerare l'IRAP determina uno svantaggio competitivo per il Mezzogiorno e per le sue imprese, oltre

cominciamo a ripristinare uno strumento che, in qualche modo, gli somigli. Non è lo strumento che vogliamo, perché ancora non è un intervento risolutivo, ma certamente è uno strumento serio che ha dato risultati importanti

chiarissimo. Tra i cinque punti annunciati dal presidente Berlusconi pochi giorni fa, e sui quali ha ricevuto la fiducia, questo punto è altrettanto chiaro. Allora, non capisco perché, quando si tratta di attuare concretamente gli impegni presi anche in sede di programma elettorale votato dagli elettori, c'è un parere negativo da parte del Governo. Ad ogni buon conto, io mi adeguo alle decisioni del mio Gruppo, Futuro e Libertà per l'Italia. intervengo solo per dichiarare che io e il senatore Firrarello voteremo a favore dell'emendamento 5.1 sul credito fiscale.

pur restando nel novero degli strumenti possibili, deve essere adeguatamente valutato. Sarei dunque d'accordo nel mutare il parere nel senso di rimettermi all'Aula, ove la presentatrice

non ha funzionato, e quindi non ho potuto votare a favore dell'emendamento

di raccordarli con i dispositivi di alcune proposte di risoluzione presentate e di determinare le condizioni per evitare che su questioni fondamentali

per gli interventi fiscali sarebbe stato più utile per raccordarsi a quanto accade nella società italiana, e non solo negli schieramenti della politica italiana. Riteniamo altresì che il tema del credito d'imposta e della fiscalità di vantaggio possa, e debba, essere affrontato in maniera organica. Il segnale che il Parlamento ha dato è sufficientemente eloquente e ci consente di poter riflettere sul prosieguo degli emendamenti.

Quello che un tempo era il DPEF e oggi è la Decisione di finanza pubblica è stato già definito sia dalla relazione di maggioranza che da quella di minoranza come un documento superato, che dovrà lasciare lo spazio e il passo ad altri

La mia personale opinione è che gli interessi del Paese e la puntualità del voto sulla Decisione di finanza pubblica valgano molto di più, avuto riguardo soprattutto agli equilibri europei, alla stabilità europea, e quindi italiana, e a quei mercati che guardano con attenzione a tutti gli atti che possano consolidare o meno

dalle migliori intenzioni, sia destinata a scontrarsi con alcuni dati di fatto ormai consuetudinari nell'agire di questo Governo che alcuni precedenti interventi hanno descritto molto bene (mi riferisco in particolare all'intervento del collega Mercatali). Ci troviamo da due anni e mezzo in una situazione nella quale la possibilità di operare sulla leva fiscale per garantire situazioni imprenditoriali in una particolare congiuntura economica italiana e - dall'altra parte - l'occupazione, assai meno per garantire l'occupazione giovanile e quella femminile, è stata da questo Governo più volte enunciata ma mai tradotta, non dico in un articolato, ma neanche in una intenzione. Ci troviamo oggi di fronte all'emendamento 5.3 della collega Poli Bortone, che ho sottoscritto, che prevede - vorrei che i colleghi

Una misura minima, ma - voglio ribadirlo - forse la prima che dall'inizio di questo Governo e dall'inizio della crisi verrebbe assunta per favorire il lavoro a tempo indeterminato di ragazze e ragazzi italiani. Non devo essere io qui a citare le cifre della disoccupazione giovanile e femminile; non sono io che devo raccontare quale disperazione

è tutto lo schema di Decisione di finanza pubblica a sottoporre all'attenzione del Senato provvedimenti importanti sullo sviluppo e sulla crescita del nostro Paese. Gli emendamenti presentati dalla collega senatrice Poli Bortone

di zone a burocrazia zero. Quindi, se la maggioranza ha bisogno di chiarirsi le idee lo faccio prima.

A me farebbe comodo, dal punto di vista politico, insistere per non sospendere la seduta, anche perché abbiamo visto che c'è una trasversalità di consensi su questo tipo di discorso. Devo dire che mi è molto dispiaciuto quello che ha detto la collega Bonfrisco. Collega, qui di strumentalizzazione non c'è niente. in una situazione felice, voi vivete in un'Italia diversa. L'Italia diversa non è quella che immaginano gli ottimi colleghi della Lega Nord, che fanno benissimo il loro mestiere. L'Italia diversa

che non intendono vivere di sommerso, alle imprese che vogliono avere un corretto rapporto con la gente che vuole lavorare, alle imprese che non vogliono essere preda diteci il motivo, un solo motivo, per il quale non si debba venire incontro, prestando un minimo di attenzione, a quegli imprenditori del Sud che, pure in un contesto così difficile, desiderano ugualmente fare impresa. Cosa stiamo chiedendo? Di venire incontro, con dei piccoli sgravi fiscali, a gente che vuole semplicemente stabilire un corretto rapporto di lavoro a tempo indeterminato con giovani, uomini e donne, che non intendono impoverire il territorio meridionale, ma lo vogliono arricchire. e gli altri desiderano convergere, ragionevolmente, su questo percorso, va bene. Se dobbiamo semplicemente perdere tempo, cari colleghi, andate pure avanti come *kamikaze* con il vostro Governo: Governo: noi continueremo ad andare avanti con la gente che vuole stare insieme con noi.

non mi piacciono, al fine di trovare un punto di intesa soddisfacente sul piano dei contenuti concreti. E visto che noi siamo un movimento politico che guarda soltanto agli interessi concreti e non a logiche a logiche schematicamente politiche, chiedo di utilizzare questa fase che si è aperta. Facciamo una sospensione, troviamoci con il Governo e giungiamo ad un punto di intesa, perché è emerso chiaramente in Parlamento il favore per questo provvedimento a vantaggio del Mezzogiorno e del suo sistema imprenditoriale.

Noi siamo favorevoli alla richiesta di sospensione.

Presidente, nella mia veste di relatrice le chiedo dieci minuti di ulteriore sospensione della seduta